In data 28 agosto 2006 e` stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri degli affari esteri e della difesa «Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l’intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite» Successivamente il Governo ha avanzato la richiesta di ritirare il provvedimento medesimo, affinche´ sia esaminato dall’altro ramo del Parlamento. La Presidenza prende atto. Il provvedimento, pertanto, verra` trasmesso alla Camera dei deputati.